di questa legislatura hanno sentito la forte necessità di migliorare le condizioni di vita del Paese, in particolare dando sostegno a coloro che avevano meno, in modo da moderare uno squilibrio socio-economico che vede tante persone non arrivare a fine mese. Quando giunge un decreto-legge, questa giusta aspirazione di ogni parlamentare, spesso coadiuvata dai suggerimenti di tante categorie che si trovano in difficoltà, conduce a un proliferare di emendamenti talora non congruenti con i dettami del Il Presidente di Commissione, che in questo caso è anche relatore, deve seguire questi dettami con le inammissibilità che sono poi supervisionate dalla Presidenza del Senato.

il libretto unico di circolazione e un bando di idee per portare le grandi navi fuori dalla laguna di Venezia. Sono temi caldi, perché nei decenni passati la nostra società ha sempre sostenuto il libero mercato e, nel caso della continuità territoriale, sia navale, sia aerea, abbiamo visto che gli imprenditori cercano giustamente il guadagno, che però, in tempi critici come quello attuale, non può realizzarsi ed è lo Stato che deve intervenire sostenendo i privati per garantire il servizio pubblico. È evidente che se non c'è guadagno i privati non si muovono, ma lo è altrettanto che lo Stato non è una vacca da mungere. Nel caso della Sardegna, il senatore Floris ha evidenziato il caso di Air Italy, che ha fatto impresa, ma che, nel momento in cui non c'è stata sostenibilità economica, non ha esitato a lasciare senza lavoro centinaia di persone. Si tratta di casi diffusi in tutto il Paese. Spesso gli imprenditori prendono le sovvenzioni statali per fare impresa, ma, nel momento in cui i guadagni vengono meno, chiudono o decentrano la propria attività. È evidente che si deve trovare un equilibrio, certamente difficile, tra queste due esigenze. La proroga riguardante il libretto unico di circolazione ha portato all'attenzione problemi immani riguardanti la circolazione, che sono stati fortemente acuiti dalla pandemia. in particolare, alle revisioni e alle patenti, con oltre 350.000 giovani che attendono anche oltre un anno per poter prendere la patente, nonché i problemi connessi alle patenti nautiche, dei rimorchi e dei mezzi agricoli.

al ritiro di numerosi emendamenti), di modo che possano essere rapidamente attuati. Il tema delle grandi navi nella laguna di Venezia è un problema immenso, perché le grandi navi hanno un pescaggio elevato e per adeguare i fondali sono stati scavati artificialmente vari canali per giungere sia in centro città, sia al porto di Marghera. Lo scavo dei canali modifica le dinamiche della laguna, sottesa di un equilibrio precario per le mutate condizioni dinamiche che ne hanno visto la nascita e l'evoluzione. Il passaggio delle navi più grandi genera correnti più intense, le quali asportano le quali asportano sedimenti, come ci è stato mostrato, sul bordo del canale dei Petroli. È evidente che erodere sedimenti all'interno dei canali può condurre allo scalzamento delle fondamenta degli edifici, con conseguenze critiche per la stabilità di questi Anche in questo caso, è necessario trovare un equilibrio tra la necessità di garantire l'arrivo dei turisti, che costituiscono una linfa vitale per l'economia cittadina, e la preservazione dell'ecosistema. Credo che l'attenzione vada posta in un'ottica di lungo termine. Le decisioni politiche troppo spesso sono legate al consenso immediato, mentre si dovrebbe volare alti e garantire la sostenibilità di un bene o di un ecosistema. Dispiacciono enormemente i giudizi del senatore De Falco, che ha criticato la decisione della 5a Commissione, quando è evidente che i suoi emendamenti, che chiedevano di procedere con la valutazione dei progetti esistenti (in pratica, solamente il progetto Duferco-De Piccoli), com'è stato evidenziato in Commissione, anche con documenti scritti a disposizione dei commissari, avrebbero certamente avuto implicazioni economiche, e non di poco conto. Ricordo - a chi non conosca il progetto - che si tratta di un porto subito fuori dalla bocca di Lido, addossato alla sponda Nord, che ha avuto un *iter* controverso. Il progetto non ha visto una gara, non ha avuto evidenza pubblica e soprattutto prevede importi preliminari di circa 140 milioni, con compensi superiori ai 5 milioni di euro; non rispetta dunque le regole dei contratti né quelle europee. Ha avuto inoltre il parere contrario sia del comitato per Venezia sia dei Comuni su cui insiste, incluso quello di Venezia. Condivido con De Falco che, comunque ci si muova a Venezia, si ledono interessi e si aprono i fuochi incrociati per bloccare questo o quel progetto. però che il ministro Giovannini - che ringrazio per aver individuato Venezia come uno dei primi temi da affrontare - abbia fatto benissimo a bandire un concorso di idee per trovare la soluzione. Ricordo che era un'iniziativa presa già dal ministro Toninelli, che aveva condotto all'individuazione di tre soluzioni fuori laguna, *iter* però interrotto dal termine del Governo Conte I. Dunque, se il progetto Duferco è valido, potrà essere ripresentato seguendo un *iter* trasparente e cristallino, che potrà eventualmente condurre alla sua approvazione. Dati i molteplici interessi, condivido perfettamente quanto esplicitato dal senatore Margiotta, ovvero che per il concorso di idee sia indispensabile individuare una commissione giudicatrice fatta da professionisti di altissimo profilo e non invischiati nel contesto locale. Troppo spesso abbiamo visto come Venezia e le opere per salvaguardarla siano state al centro di malaffare e truffe. Ricordo che, quando siamo giunti al Governo noi del MoVimento 5 Stelle, il Mose non era stato completato, benché mancasse solamente un 5 per cento per il completamento dell'opera. Oggigiorno forse si potrebbero trovare soluzioni alternative e meno impattanti sull'ecosistema della laguna, ma intanto è stato avviato e protegge Venezia dalle maree eccezionali, sempre che chi è preposto alle decisioni lo faccia con prontezza.

che l'importante dibattito che c'è stato in Commissione e la produzione di emendamenti non ostruzionistici, ma di merito e rispondenti a esigenze reali che si avvertono nel Paese, abbiamo potuto arricchire tutti noi in termini di competenze e di conoscenze. Vorrei sottolineare che anche le proroghe, quando non si è stati capaci di completare l'*iter* o di dare soluzione alle questioni, sono uno strumento importante per non aggravare le difficoltà dei soggetti interessati. Questo è il lavoro che abbiamo fatto. Tanti emendamenti sono stati presentati e condivisi, ma purtroppo non andranno in discussione e non sarà possibile approvarli, perché sono stati dichiarati inammissibili. Quegli emendamenti però, come dicevo in precedenza, hanno segnalato esigenze reali, a cui bisogna dare soluzioni.

fare in modo che ci siano i tempi per migliorare il provvedimento alla Camera dei deputati e comunque occorre impegnarsi per trovare uno strumento con cui poter dare soddisfazione al grande lavoro che è stato fatto. Grazie ancora e buon lavoro a tutti noi.

gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 2.8 (testo 2), 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11,

favorevole

Per ragioni di coordinamento normativo, atteso che il contenuto delle proposte emendative 3.0.10 (già 3.29), 3.0.3

«impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie a garantire il coinvolgimento delle associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,

Un costo verrebbe a configurarsi solo dopo l'eventuale approvazione di uno dei progetti (non ve n'è uno solo) che sono in questo momento presenti ad uno stadio avanzato. Ho raccolto 15 firme dei colleghi e chiedo che sia messo comunque ai voti, perché l'interesse nazionale è stato anche illustrato dal ministro Franceschini ed è quello di far allontanare al più presto le navi dalla laguna veneta. Con l'articolo 3, che è contenuto nel decreto-legge n. 45, non abbiamo certezza che tra cento anni le navi non siano ancora lì. Con l'emendamento 3.1, invece, si chiede sostanzialmente di esaminare almeno i progetti esistenti e non buttare tutto il lavoro che è stato fatto, senza neanche esaminarlo. L'esame non comporta la spesa: questo è il punto.

del Governo, quando è arrivato in Commissione questo decreto-legge recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, che ci apprestiamo a convertire, abbiamo pensato che potesse rappresentare un'occasione per la trattazione seria di queste tematiche e abbiamo discusso e lavorato per dare un senso alla normativa proposta. non vi dico nulla, ma cortesemente accomodatevi fuori dall'Aula. Prego, senatrice. VONO *(IV-PSI)*. Devo dire, però, che il fatto che la maggior parte degli emendamenti presentati e su cui spesso si è trovato anche l'accordo della maggioranza dei Commissari voglio ribadire che non erano emendamenti bandiera per i nostri partiti politici di appartenenza, ma utili e necessari ai cittadini e alle imprese che, fiduciosi, ci avevano chiesto di intervenire) siano stati dichiarati quali improponibili, quali bocciati, perché non rispettosi dell'invarianza finanziaria, e quali (pochi) rimodulati, non ha sicuramente conferito al documento finale l'efficacia che avrebbe potuto avere con il loro accoglimento. Purtroppo e mi riferisco al Presidente di Commissione - rileggendo le relazioni tecniche ad alcuni emendamenti di puro carattere ordinamentale, ho potuto rilevare - certamente è una mia opinione personale, che esprimo comunque come Vice Presidente di Commissione - un eccessivo e forse anche discutibile rigorismo discrezionale, che non ha valutato e tenuto in debito conto le urgenze determinate dal periodo che stiamo vivendo di forte e aggravata crisi economica, rendendo il decreto-legge insufficiente sotto vari punti di vista, che non stiamo qui a discutere, perché sono stati ben esplicitati negli interventi della discussione generale di ieri, che ne hanno evidenziato con chiarezza le criticità. Tuttavia ci è stato rappresentato un lavoro del Governo su un imminente decreto oggetto dell'odierno Consiglio dei ministri, che dovrebbe riguardare in modo quasi esclusivo proroghe di alcuni termini che rientrano nella materia degli emendamenti esclusi e che quindi dovrebbe accogliere molte delle istanze rimaste inevase. Si tratta - lo ripeto - di richieste avanzate dai cittadini e dalle imprese, di cui siamo i legittimi rappresentanti, proprio sulla base della nostra democrazia costituzionale, ritenendo - ne siamo sicuri - che questo nuovo decreto non lasci - come accaduto per quello di oggi - solo l'amaro in bocca.

sempre presente in Commissione a dare il giusto supporto, con collaborazione e aperto confronto, e del lavoro svolto da tutti i colleghi; confidando nell'azione e concreta di interventi validi e fondamentali, in un settore così importante e strategico come quello dei trasporti; e augurandoci che, usciti dalla fase dei provvedimenti di emergenza, noi parlamentari e la Commissione cui appartengo possiamo finalmente svolgere in modo esaustivo e incisivo il nostro ruolo nostro ruolo di rappresentanti dei cittadini, ma ancor più di legislatori (che è la nostra funzione principale in Parlamento, sempre e comunque);

Signor Presidente, questo decreto-legge è stato chiamato impropriamente "decreto Venezia". Esso in realtà tocca argomenti che hanno grande rilevanza pratica: mi riferisco all'articolo 1, nel quale si parla delle disposizioni in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, e all'articolo 2, che reca disposizioni e misure urgenti in materia di documento unico di circolazione. Nella disciplina del trasporto marittimo, in particolare, la priorità per Fratelli d'Italia è che sia garantito con continuità il servizio di trasporto con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti. Si tratta di collegamenti di interesse nazionale, la cui continuità è essenziale per garantire il diritto alla libertà di movimento dei cittadini. Questo vale sia per le tratte restituite al libero mercato, in quanto ritenute contendibili da diversi operatori marittimi, sia per quelle a regime di servizio pubblico, per le quali hanno preso avvio le procedure di gara. Signor Presidente, sono proprio queste procedure che ci preoccupano, perché secondo molti operatori contengono clausole suscettibili di essere impugnate. Abbiamo timore per i tempi e soprattutto temiamo che queste circostanze possano ripercuotersi sul servizio offerto ai cittadini. Fratelli d'Italia sarà vigile e attenta su tali aspetti. Porre a gara un servizio di continuità territoriale non è un gioco politico da sfruttare elettoralmente; i servizi di continuità territoriale sono essenziali.

a intervenire. Indispensabile è l'attenzione che chiediamo alla tutela del lavoro e dei lavoratori del settore, già abbastanza gravati dalla crisi. L'articolo 2, che cita la proroga del documento unico, in realtà avrebbe dovuto affrontare seriamente l'emergenza, che coinvolge un numero elevatissimo di giovani, che non riescono a ottenere in tempi ragionevoli la patente di guida indispensabile per il lavoro, la Carta infatti assurdo, quanto irragionevole, che a causa di questa problematicità moltissime aziende che hanno bisogno di lavoratori con determinate patenti non stiano assumendo. Moltissime società sono alla ricerca di lavoratori muniti di patenti superiori e ci sono tante persone che materialmente non riescono a conseguire le certificazioni richieste. Ci sono, per esempio, aziende impegnate nella raccolta di rifiuti urbani, che noi di Fratelli d'Italia abbiamo contattato e con le quali abbiamo provato a interagire, che chiedono di rivedere tutta la normativa vigente. Già da qualche anno abbiamo provato a chiederlo in Commissione, ma purtroppo, ricollegandomi a quanto detto da autorevoli colleghi della maggioranza, il ruolo delle Commissioni è svilito

Rispetto al 2010 si sono ridotti addirittura del 48 per cento i candidati al conseguimento di patente C, per una serie di fattori (alti costi, bassissima percentuale di candidati che superano l'esame e tempi molto lunghi per il conseguimento). Abbiamo proposto in via emendativa,

la possibilità di guidare questi veicoli di massa alla fine non superiori alle sette tonnellate e ciò per favorire un rilancio dell'economia, per consentire in qualche modo qualche modo a queste aziende di poter assumere in maniera più facile in un momento di grande crisi. Ci è stato risposto che questo emendamento non era ammissibile, come se fosse invece ammissibile che lo Stato paralizzi l'offerta di lavoro in un momento così critico per la nostra economia. Ci sono poi casi incredibili di tanti cittadini che versano soldi al Ministero per sostenere due prove d'esame (quiz e guida) da svolgere entro sei mesi a causa delle chiusure del Governo e della carenze di personale ormai endemica nelle motorizzazioni, non riescono a concludere in tempo il percorso semestrale previsto. Quindi si iscrivono, ma lo Stato purtroppo non li mette in condizioni di sostenere l'esame e perdono addirittura i soldi. Il caos delle motorizzazioni - sappiamo benissimo che gli uffici preposti non riesco nemmeno a a smaltire gli arretrati - è ai limiti dello scandalo. Avremmo voluto contribuire a mettere un po' di ordine nel caos, ma lo svuotamento del nostro ruolo nelle Commissioni non ce lo ha oggettivamente consentito. rispetto all'articolo 3 in cui si parla di Venezia, basterebbero le parole di un poeta per spiegare la nostra posizione: «(...) le stelle sbiadiscono di invidia vedendo emergere dalla nebbia gli incanti di Venezia». Questa bellezza dobbiamo preservarla e sarebbe stato facile farlo. Non servono un concorso, grandi iniziative pubblicitarie,

basta difendere la storia, l'identità e le caratteristiche che fanno di Venezia una delle città più belle, indimenticabili e visitate di tutto il Pianeta. Avremmo voluto dare di più. In parte alcune nostre idee, alcuni nostri consigli sono stati accolti e alcuni nostri emendamenti inseriti nel decreto che verrà, per cui la nostra sarà un'astensione responsabile, anche se, ripeto, avremmo voluto dare di più.

le pubbliche amministrazioni, ha rallentato gli *iter* autorizzativi e, quindi, sarebbe stato assolutamente impensabile e irresponsabile non prendere atto che, anche per le questioni relative ai trasporti, ciò non stesse accadendo. Di conseguenza, con questo provvedimento del Governo

incentrata sulle grandi navi a Venezia, che è una questione annosa. Venezia è la città di tutti. Quando parliamo di Venezia, tutti ci sentiamo veneziani, non solo chi, come il sottoscritto, è nato e risiede in quella meravigliosa realtà, ma tutti gli abitanti del mondo. Non a caso, quando cade uno spillo a Venezia, ne parlano i comitati UNESCO, i comitati

la complessità. Presidente, credo che il Governo e il Parlamento abbiamo il compito di ascoltare tutti e poi decidere. Bisogna ascoltare i comitati ambientalisti, che storicamente hanno combattuto delle nobilissime battaglie per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, laguna, ma anche le categorie e i vari mondi dell'economia, che attraverso il porto hanno generato, generano e devono continuare a generare lavoro anche nei prossimi anni. La politica, però, non deve rappresentare solo un interesse. Qui non dobbiamo rappresentare la decisione del comitato o l'interesse o l'interesse legittimo della singola categoria. La politica ha il compito di operare la migliore sintesi all'interno di questa complessità. Presidente, crediamo che la decisione debba muoversi all'interno di due polarità, secondo noi, irrinunciabili. La prima è che Venezia senza un porto non si può neppure immaginare. Venezia è nata con il suo porto; Venezia ha sempre vissuto l'Adriatico, quel braccio di mare del Mediterraneo, non come difesa o come separazione, ma come ponte ma come ponte non solamente dei commerci. La Serenissima è stata non solo regina dei commerci, ma anche della politica, delle relazioni, della cultura e ha fatto della differenza la propria ricchezza. Era talmente consapevole della grandezza della propria identità da potersi permettere di dialogare con culture diverse. Ha inoltre, attraverso la diversità di queste culture la sua identità perché Venezia ha accolto, come ho già avuto modo di ribadire in quest'Aula, culture e mondi spesso anche minoritari che venivano cacciati come i greco-ortodossi, gli armeni e gli ebrei. Li ha vissuti come ricchezza e come parte della propria identità. Quando parliamo di Venezia, parliamo dell'esempio per il futuro di ciò che deve essere la nostra nazione. È il ponte dell'Europa nei confronti delle politiche del Mediterraneo,

che non c'è mai stato nella storia della Serenissima. Ora siamo in presenza di navi con stazza lorda di 150.000 tonnellate, con lunghezza che supera i 350 metri. Sappiamo, perché in quest'Aula dobbiamo essere innanzitutto che oggi nella laguna non possono entrare le navi con stazza lorda superiore a 96.000 tonnellate. Voglio, però, anche ricordare gli episodi della nave che ha cagionato, nel 2019, quell'incidente che è stato mostrato a tutto il mondo, nella banchina di San Basilio, e della

erano all'interno delle 96.000 tonnellate, ma erano di 292 metri: quindi, dei grattacieli veri e propri, che ancora oggi entrano nella nostra laguna. Ne deriva che il gigantismo navale non è accettabile nella nostra laguna, perché va contro la sua stessa identità. Non stiamo dicendo cose del tutto innovative, perché il PAT, il piano dell'assetto territoriale votato dal Comune di Venezia e dall'amministrazione comunale di Venezia nel 2012, definisce già il concetto di fondo di classe Venezia per le navi, dicendo che devono entrare in laguna quelle compatibili con l'ecosistema. Ma l'ecosistema è anche l'ecosistema economico, perché se noi non consideriamo seriamente questa questione creiamo il miglior alibi per chi, semplicemente, vuole chiudere il porto. Se, invece, realizziamo un porto sostenibile, come richiede il nuovo concetto di sostenibilità, creiamo anche le condizioni di sviluppo economico del porto.

perché sono assolutamente migliorativi. Ritorno alla classe Venezia di cui prima, perché non basta la stazza lorda, ma bisogna parlare anche di dislocamento.

perché è stato siglato da tempo un accordo di programma tra l'autorità portuale e gli enti locali in questa direzione. Noi volevamo fosse riconosciuto a livello di decreto e abbiamo voluto votarlo in Commissione ambiente. Quindi, quello rimane una pietra miliare per le politiche e le decisioni future.

perché non possiamo più prenderci in giro. Dobbiamo andare a verificare immediatamente la possibilità di realizzare queste opere. Da ultimo, la commissione valutatrice deve essere di alto profilo, perché Venezia è Venezia, perché la laguna è la laguna. Quindi, indichiamo al Governo, all'interno del decreto, questa decisione, secondo noi di fondo, già ripresa all'interno della Commissione ambiente. Infine, naturalmente, no allo scavo di nuovi canali. Vittorio Emanuele è stato oggetto di dibattito nella Commissione. Abbiamo trovato un giusto equilibrio perché certamente l'apertura del nuovo canale Vittorio Emanuele, chiuso di fatto da tempo dopo l'apertura del canale dei petroli,

il decreto che ci accingiamo a convertire ha rappresentato, nell'ambito dell'*iter* in Commissione, un'occasione certamente proficua per l'ascolto di professionisti, operatori e organizzazioni del settore, che come sempre hanno dato un apporto qualificato e significativo per consentirci di integrare e migliorare l'intervento. In questo senso, il lavoro in Commissione è stato certamente articolato e abbiamo condiviso con i colleghi che il tema dei trasporti, e più in generale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, si conferma come cruciale per il presente e per il futuro del Paese. va fatta una riflessione: molti emendamenti sono stati presentati, naturalmente condivisi da più forze politiche, quindi con una forte convergenza, ma tutto ciò non ha permesso e questa credo sia la prima riflessione che va fatta con il Governo. Infatti, se il ruolo dell'Assemblea e delle Commissioni

Se guardiamo al solo contenuto del provvedimento, infatti, anche all'esito della fase emendativa, non possiamo negare che avremmo voluto fare di più sia per le problematiche connesse alla pandemia, sia più in generale per altri aspetti per nulla irrilevanti. quindi, su due articoli ci siamo mossi solo su delle proroghe, quindi importanti ma poco sostanziali, mentre sull'articolo 3, dove invece abbiamo trattato la questione Venezia, va fatta una riflessione molto molto importante. Venezia è un patrimonio mondiale dell'umanità e quindi credo che l'accelerazione e l'azione del decreto verso un concorso di idee siano elementi di fondamentale importanza e in questo caso la convergenza è determinante e imprescindibile.

analizzate da professionisti di livello assoluto. Credo che questo possa essere un altro emblema della grande capacità di questo Paese

in merito alle riflessioni suddette, non possiamo negare che, dove interviene, il provvedimento è certamente utile. Credo che la velocità e la pragmaticità con cui aggiungeremo a questo altri interventi, a partire ovviamente dal PNRR, determineranno l'efficacia di un'azione più completa e utile al Paese, un'azione che consenta di tenere insieme, in modo virtuoso e sostenibile, economia, turismo, salvaguardia dei beni culturali e crescita;

Signor Presidente, siamo riusciti con l'Aula quasi deserta ad avere silenzio; questo è fondamentale.

posto dalla Commissione bilancio, per la quale condivido abbastanza le parole del senatore Coltorti; non c'è una criminalizzazione nei confronti del suo lavoro, ci mancherebbe altro.

cui in qualche modo la Commissione bilancio dovrebbe necessariamente tener conto perché la contenutistica, indipendentemente dall'aspetto di bilancio che è fondamentale, è essenziale per una risposta che il cittadino e il sistema vogliono portare avanti.

Più volte ho tentato, anche personalmente, come parlamentare della Repubblica, di spiegare la necessità che questa azienda se vuol andare avanti, deve guardarsi intorno,

nell'affrontare la questione di chi fa prima l'esame rispetto al numero dei fogli rosa, che le piccole e le grandi agenzie che si occupano di tali questioni portano all'attenzione della motorizzazione della Provincia. Ce ne sono alcune che avvantaggiano il grande numero ed altre che avvantaggiano il piccolo; a mio avviso bisogna dare una linea e sono convinto che potremmo anche trovare una soluzione. Il tema più politico del decreto-legge è Venezia, è Venezia, uno degli argomenti più delicati da affrontare. Devo dire che sono anche un po' soddisfatto della dichiarazione che ha fatto il presidente Coltorti:

piaciuto perché in questa legislatura sostituisco una grande persona che sul Mose ci ha sempre messo la faccia e si è speso: era il suo predecessore alla guida della Commissione infrastrutture e trasporti, il senatore Altero Matteoli che è stato additato non so quante volte per una scelta di questo tipo. Se oggi Venezia è salva - ho sentito ieri una descrizione

Anche l'antropizzazione di Venezia è stato l'elemento che ha costruito quella città: se oggi c'è Venezia, è perché qualcuno l'ha realizzata; se oggi c'è Venezia, è perché qualcuno ha scavato i canali i canali e perché qualcuno l'ha resa una città importante dal punto di vista commerciale. Voglio ricordare che essere Repubblica marinara all'epoca non voleva dire: aspettiamo che arrivino i turisti da Pisa

altre importanti strutture ricettive che aspettavano i turisti o ristoranti come il Do Forni per andare a pranzo o a cena. Non ho questo ricordo della storia della fondazione della città di Venezia. Credo che questo ricordo non lo abbiano nemmeno i 13.000 13.000 addetti del Porto di Marghera. Se vogliamo levare le navi commerciali, le navi passeggeri, il porto, le raffinerie e qualsiasi cosa, facciamo tutto da qualche parte (non si sa esattamente dove),

ammazziamo il secondo, terzo o quarto - a seconda delle tipologie di prodotto lì utilizzate - porto italiano; uccidiamo la storia d'Italia con la Venezia commerciale; massacriamo la prospettiva industriale del Nord-Est italiano; chiudiamo tutto tutti a casa perché saremo tutti pubblici dipendenti, lavoreremo tutti nella scuola, lavoreremo tutti nei palazzi del potere. C'è una cosa che forse sfugge: ci sarebbero anche le imprese in Italia. Sono imprese che lavorano, che fanno produzione, che trasportano, che danno una prospettiva. Noi siamo consapevoli che le navi non debbano passare dal canale della Giudecca, ovviamente, perché prima o poi qualcuna

follia. Su questo noi saremo vigili; ho sentito che il collega Ruspandini sarà vigile anche lui, e mi fa piacere, perché porta sempre un grande contributo alla Commissione. Noi saremo vigili e fattivi come parte di questo Governo perché vorremo intanto che quella Commissione, quel gruppo di lavoro, non si trastulli per quattro o cinque anni. Anzi, qui bisogna parlare di settimane: dobbiamo fare in modo che il Governo assegni, attraverso il Ministro, il Vice ministro e tutta l'organizzazione politica che questa maggioranza sostiene, degli obiettivi quotidiani o settimanali *(Applausi)*, perché vogliamo delle risposte subito.

Oggettivamente gli insulani rischiavano di vedersi privati del loro diritto di essere collegati con il Continente per i ritardi che ci sono stati di chi doveva bandire le gare per tempo, e non lo ha fatto nei tempi dovuti. Ora, abbiamo messo una piccola pezza e speriamo che, nel giro di poche settimane, si arrivi alla conclusione delle gare così da poter garantire in maniera continuata i diritti di tutti.

ha voluto il coinvolgimento delle associazioni di categoria, sempre a beneficio dei consumatori, dei clienti. Si è poi parlato - e non posso esimermi neanche io dal fare un breve passaggio - della parte che riguarda Venezia,

nulla ci "azzecca"; anzi, una città che vive prettamente di turismo si è vista privata di questa importante entrata economica. Una città che vede un calo demografico, come abbiamo detto anche ieri: da 150.000 a 50.000 persone in pochi decenni.

dobbiamo anche chiederci di cosa deve vivere Venezia a questo punto. I turisti li vogliamo o no a Venezia? È una scriminante che dobbiamo tenere ben presente; non possiamo esimerci dal porci questa domanda. Dobbiamo

Andiamo a parlare del personale delle motorizzazioni, che manca; delle regole per l'utilizzo della targa prova; delle patenti nautiche; di un'incentivazione seria per il rinnovo del parco autoveicoli.

stiamo parlando di un provvedimento che a prima vista risulta piccolo e scarno, perché è composto da pochi articoli, ma in realtà essi esprimono un alto contenuto. parlando, innanzitutto, di continuità marittima per le isole, come Sardegna, Sicilia e Tremiti. Si tratta di un servizio indispensabile per gli isolani, che per il MoVimento 5 Stelle è garanzia del diritto di mobilità, sia per le persone che per le merci. necessario discuterne oggi, affinché si evitino interruzioni del servizio di continuità marittima. È una piccola proroga, che di fatto permetterà di concludere le procedure già bandite per la concessione e che dà garanzia dei servizi di continuità marittima per le nostre isole, minori e maggiori.

uno strumento di semplificazione, che accorpa le procedure di immatricolazione e di trasferimento di proprietà. Il MoVimento 5 Stelle accoglie con favore le procedure telematiche di semplificazione. Ma ciò che vorrei raccomandare in quest'Aula, oggi, al Governo, è la necessità di una più assidua e leale interlocuzione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Si tratta dei principali attori di questo processo telematico, che hanno rappresentato a noi parlamentari, in Commissione, la necessità di maggiore coinvolgimento sugli aspetti operativi, che poi vengono essenzialmente rimessi a loro e alla loro intermediazione. Questa è una raccomandazione accurata che il Gruppo MoVimento 5 Stelle oggi vuole rimarcare. Infine, parliamo della laguna di Venezia e della necessità di preservare e tutelare quel fantastico ecosistema nella sua interezza. decreto-legge sancisce finalmente l'avvio di un processo, che venne definito, nel 2012, attraverso un decreto ministeriale, il cosiddetto decreto Clini-Passera, e che sancì l'estromissione del passaggio delle grandi navi dal canale di San Marco. Permettetemi di dire che il decreto-legge in discussione oggi fa molto di più e, infatti, prevede l'individuazione di punti di attracco al di fuori dalle acque della laguna, per le navi di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, quindi le grandi navi. Ciò significa che si va oltre le 78 paratoie del Mose e si va lontano da Marghera. Da oggi ha inizio un processo di eliminazione delle grandi navi dalla laguna e questo ci rende fiduciosi che il percorso andrà a buon fine. deve essere messa nelle condizioni di poter mantenere quell'equilibrio, molto delicato e sensibile, che la caratterizza e, dunque, l'uomo e la politica hanno il preciso dovere di tutelare questo equilibrio lagunare, per tutelare la laguna stessa. Gli stessi scavi e le operazioni di dragaggio dei canali devono avere come priorità il ripristino della morfologia originaria della laguna, che già risente negativamente degli effetti delle acque del mare, che entrano attraverso le bocche di porto, nel canale dei petroli. Colleghi, il contesto di emergenza climatica che viviamo, con l'innalzamento delle acque marine, con il fenomeno dell'erosione costiera e con tutti gli effetti catastrofici ad essa legati, non può e non deve lasciarci indifferenti. Così come non possiamo e non dobbiamo restare impassibili dinanzi alle criticità di ordine ambientale e paesaggistico, relative ad un patrimonio unico al mondo, come quello gelosamente custodito a Venezia. Alcuni colleghi di altre forze politiche hanno argomentato il tema, evidenziando l'essenzialità dell'aspetto economico derivante dall'indotto turistico crocieristico su Venezia. Questo è verissimo, ma mi chiedo fino a che punto l'aspetto della tutela ambientale possa cedere il passo a quello della tutela economica; fino a che punto fino a che punto possa continuare ad esistere un'economia là dove la natura subisce abusi. Quello che ci aspettiamo è il raggiungimento di un giusto equilibrio tra questi due aspetti; diversamente, cari colleghi, dove perisce la natura l'indotto economico muore.

alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

il ritiro dei contingenti NATO e degli Stati Uniti dell'Afghanistan è ormai imminente. È una missione alla quale l'Italia ha contribuito dall'inizio, e quindi dal 2001. Dopo l'attentato alle Torri gemelle per la prima volta stato utilizzato l'articolo 5 del Trattato NATO, secondo il quale, quando viene colpito un Paese dell'Alleanza, anche gli altri Paesi sono chiamati a intervenire. L'obiettivo era contrastare il terrorismo di al Qaeda. Abbiamo partecipato con ruoli rilevanti nella catena di comando della missione e abbiamo avuto da subito, appena si è un po' stabilizzato il Paese, la responsabilità del PRT di Herat, cioè della regione ovest.

sono morti lì, sul suolo afghano: un sacrificio e un prezzo altissimo che non dobbiamo dimenticare. Il Ministro della difesa ha avuto modo di dichiarare che il nostro obiettivo è conservare i risultati fin qui conseguiti; obiettivo sul quale sono certa che anche lei concorda. Tra i risultati conseguiti c'è indubbiamente stato un miglioramento della condizione di vita delle donne. Nel regime dei talebani le bambine non andavano a scuola e neanche molti bambini; solo 900.000 ragazzini

Dei passi in avanti sono stati fatti, in una situazione che - ripeto - rimane ancora complicatissima, con le spose bambine e con le lapidazioni. Ho incontrato alcune volte le rappresentanti delle donne afghane, donne davvero lucide e coraggiose, cui preoccupazione, nel momento in cui il contingente internazionale andrà via, è che tutto torni come prima. Da tempo sono in corso delle trattative fra rappresentanti del Governo statunitense e il Governo afghano, i talebani,

Signora Presidente, ringrazio la senatrice Pinotti. L'Afghanistan si trova oggi a uno snodo cruciale della sua storia. Restituire stabilità al Paese e creare le condizioni per la riconciliazione nazionale sono obiettivi per i quali per la prima volta si è aperta una finestra. Questo percorso, certamente complesso, dovrà consentire di preservare i fondamentali progressi compiuti negli anni dal Paese, anche grazie all'Italia come ha detto la senatrice interrogante - specialmente nella protezione dei diritti di donne, bambini e minoranze. È un aspetto per noi imprescindibile, come ho avuto modo di sottolineare anche alla ministeriale NATO dello scorso 14 aprile. Una nuova generazione di cittadine e cittadini afghani, cresciuti negli ultimi venti anni, auspica un futuro in cui i diritti umani e le libertà fondamentali siano rispettati. Le loro voci meritano ascolto in sede di negoziato. Il loro ruolo nella società deve essere tutelato dopo la conclusione dell'accordo di pace. Il mese scorso, nel dibattito dedicato all'Afghanistan nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, abbiamo espresso l'auspicio che le Nazioni Unite possano svolgere un ruolo di primo piano nei negoziati di pace intra-afghani. Ciò offrirebbe una rassicurazione ulteriore sull'attenzione al tema dell'eguaglianza di genere nei futuri sviluppi del processo. Il nostro Paese sin dall'inizio ha ispirato la propria azione in Afghanistan a questi principi. Negli ultimi due decenni, con un attento monitoraggio del rispetto dei diritti umani, abbiamo esercitato, assieme a *partner* e alleati, pressioni diplomatiche sulle autorità locali per indurle a iniziative più energiche in questo settore cruciale. la cooperazione allo sviluppo ha finanziato progetti per promuovere uguaglianza di genere e salute riproduttiva, sviluppare la micro-imprenditoria femminile, prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere, ridurre la mortalità materna e infantile. I nostri progetti di cooperazione continueranno. In occasione della più recente sessione di revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, l'Italia ha rivolto alle autorità di Kabul specifiche raccomandazioni in materia di diritti delle donne e dei bambini. La dimensione di genere e il rispetto dei diritti fondamentali hanno costituito tematiche trasversali anche del nostro impegno nel sostenere e formare le Forze armate e di polizia dell'Afghanistan. Nel quartier generale a guida italiana di Herat è stata introdotta la figura del consigliere del comandante per le questioni di genere, per l'attuazione della risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza, che esorta a incrementare la partecipazione delle donne e a integrare le prospettive di genere negli sforzi delle Nazioni Unite in materia di pace e sicurezza. In vista della conclusione della missione "Resolute Support", il Ministero della difesa ha assicurato la disponibilità a esplorare da subito forme di collaborazione con le autorità afghane per continuare, ove possibile, queste attività e per questo vorrei ringraziare il ministro della difesa Lorenzo Guerini. In conclusione, il ruolo dell'Italia e degli alleati in Afghanistan non si esaurirà con la missione NATO. Resteremo impegnati a monitorare e a mettere in atto ogni opportuna azione affinché le prossime tappe dei negoziati di pace intra-afghani pongano al centro il tema delle conquiste politiche e sociali degli ultimi due decenni, a partire dai diritti delle donne e delle minoranze etnico-religiose. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per permettere all'Afghanistan di tornare a crescere in un clima democratico e di pace.

Lei ha detto che l'Afghanistan è a un nodo cruciale della sua storia e penso che, per il ruolo che abbiamo avuto e per i legami di profonda amicizia che quel popolo sente nei nostri confronti, dobbiamo essere impegnati al massimo a non lasciarli soli, a non tornare indietro. Ha ricordato che abbiamo formato una parte significativa delle Forze armate e delle Forze di polizia dell'Afghanistan. Molte donne ne fanno parte e ha ricordato il nostro lavoro. Pensate che nella provincia di Herat abbiamo costruito insieme alla cooperazione un campo, un carcere femminile, che sembrerebbe una cosa negativa, ma per le donne afghane picchiate, torturate e violentate e per le bambine che sono scappate da matrimoni è stato, invece, un rifugio; una sorta di casa per le donne maltrattate e non un carcere femminile.

fare la stessa cosa e aiutarle, come abbiamo fatto in quel momento.

Considerato che la *United Nations relief* and works *Agency* for palestine refugees (UNRWA) ha tra i suoi scopi il sostegno e la promozione di iniziative a favore dei rifugiati palestinesi; considerato, inoltre, che il Governo italiano ha recentemente incrementato il Fondo iniziale destinato all'Agenzia stessa delle Nazioni Unite per un importo pari a due milioni di euro, raggiungendo così l'importo stanziato di euro; visto che, tra le lodevoli iniziative poste in essere dall'Agenzia, vi è anche la diffusione dell'insegnamento e della formazione; visto, inoltre, che tra queste iniziative vi è la pubblicazione di materiale scolastico distribuito tra gli studenti palestinesi, con stupore abbiamo appreso che tra queste pubblicazioni ve ne sono numerosi che contemplano l'odio verso Israele ed esaltano la *jihad*, come peraltro evidenziato nei giorni scorsi da un articolo sul sito formiche.net. Signor Ministro, le chiediamo se innanzitutto è a conoscenza

Inoltre, vogliamo sapere le modalità di monitoraggio che il nostro Paese, quale membro dell'Advisory Commission UNRWA, pone in essere affinché non si abbia più a ripetere una tale circostanza come ella potrà certificare certamente - è in palese violazione dei principi cardine contenuti nella nostra Carta costituzionale.

È in questa prospettiva che si inserisce il contributo della cooperazione italiana all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, che opera in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e striscia di Gaza. Sono aree prioritarie per l'Italia, tanto più in una fase resa ancor più drammatica dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni al movimento internazionale di beni e personale umanitario. Vengo al quesito specifico. Sul tema dei libri di testo utilizzati nelle scuole gestite dall'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, tema sollevato dai rapporti pubblicati da Impact-SE, organizzazione *no profit* basata in Israele, vorrei assicurare che il Governo segue la questione con particolare attenzione, anche nel quadro del dialogo tra Agenzia e donatori. In quanto membro della Commissione consultiva dell'Agenzia, l'Italia partecipa, per il tramite del Consolato generale a Gerusalemme, alle varie riunioni di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Nel corso degli ultimi incontri l'Agenzia ha fornito chiarimenti puntuali proprio in risposta alla richiesta di massima trasparenza avanzata dai donatori, Italia inclusa, su questa vicenda. In un primo documento dello scorso gennaio, la Impact-SE aveva, infatti, criticato i messaggi, ritenuti non in linea con i valori delle Nazioni Unite, e i contenuti dei materiali utilizzati nelle scuole gestite dall'Agenzia ONU per la didattica *online* nel periodo febbraio-novembre 2020. Il vertice dell'Agenzia ha risposto con una lettera ai membri della Commissione consultiva. Nella lettera il commissario generale ha fatto presente che l'Agenzia utilizza un sistema interno di revisione permanente dei materiali scolastici. Come risultato della revisione, l'Agenzia aveva deciso di rimuovere i materiali didattici ritenuti effettivamente non in linea con gli standard delle Nazioni Unite. Successivamente, a febbraio, Impact-SE ha pubblicato un secondo rapporto in cui punta il dito anche contro i materiali di autoapprendimento utilizzati nel periodo novembre 2020-gennaio 2021. Al fine di non lasciare dubbi circa la politica di tolleranza zero verso ogni atto di discriminazione e di incitamento alla violenza, l'Agenzia ha risposto a questo secondo rapporto sospendendo in via precauzionale la piattaforma allora utilizzata, contenente i materiali didattici in questione al fine di garantire un ulteriore approfondito esame ad opera di un organo neutrale di valutazione, appositamente creato. Il 19 aprile, nel corso di un incontro con i membri della Commissione consultiva, a cui l'Italia ha partecipato, l'Agenzia ha annunciato la conclusione del processo di revisione e la decisione di adottare una nuova piattaforma per i materiali di autoapprendimento. Anche grazie a questa piattaforma, d'ora in avanti, qualsiasi materiale *online* utilizzato nelle scuole gestite dalle Nazioni Unite, dove la modalità di didattica a distanza è tutt'ora prevalente, dovrà superare una valutazione ancora più stringente, cui parteciperanno personalmente dirigenti dell'Agenzia al più alto livello. Questo è l'impegno preso. La Farnesina, anche per il tramite del Consolato generale d'Italia a Gerusalemme, continuerà ad esercitare un ruolo di vigilanza sulle iniziative dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, in modo da prevenire ogni discordanza fra le attività finanziate e i principi cardine della cooperazione italiana, quali la non discriminazione e il sostegno alla convivenza pacifica.

Non è questa la sede per aprire un dibattito sulle ragioni dei 5 milioni di rifugiati; non è questa la sede per dire che ci sono razzi che partono da Gaza. Non è questo il momento.

vogliamo monitorare costantemente, non vogliamo abbassare la guardia, perché l'intento non è discriminatorio, ma è ribadire la tolleranza zero verso l'odio, da chiunque esso provenga. Pertanto, la ringrazio, signor Ministro.

tra le principali e più importanti misure adottate per far fronte all'emergenza Covid-19, ha assunto un rilievo notevole, fin dai primi mesi del 2020, il cosiddetto blocco dei licenziamenti. Con questa misura si è inteso impedire alle aziende di licenziare i propri dipendenti per ragioni economiche, sia in forma collettiva, sia in forma individuale. L'obiettivo dell'allora Governo Conte-*bis* era quello di evitare che le conseguenze più crude dell'emergenza venissero addossate sulle classi lavoratrici, trasformando così una crisi sanitaria e una crisi economica addirittura in una crisi sociale. D'altro canto, sono stati molti gli interventi normativi che hanno consentito il ricorso agli ammortizzatori sociali, come la Cassa integrazione guadagni il Fondo di integrazione salariale (FIS), soprattutto al fine di supportare le aziende che maggiormente hanno risentito della diminuzione della domanda di beni e servizi e, in special modo, quelle imprese attive in settori cruciali, come il turismo e la ristorazione. Il cosiddetto decreto sostegni ha previsto la fine del blocco dei licenziamenti, con riguardo al tipo di ammortizzatore sociale a cui si fa ricorso. Il 30 giugno, infatti, termina il blocco per le imprese che usufruiscono della CIG ordinaria; per lo più sono le imprese del settore industriale. Il 31 ottobre, invece, rappresenta il termine per il blocco dei licenziamenti delle aziende beneficiarie delle 28 settimane di assegno ordinario a carico del FIS o di cassa integrazione in deroga. Signor Ministro, si apprende da sue interviste recenti che l'intenzione del Governo sarebbe quella di predisporre ritocchi alle normative per sostenere il superamento del blocco dei licenziamenti con strumenti che tengono conto del diverso andamento dei settori. premesso, vorrei chiederle quali iniziative urgenti intenda promuovere al fine di rilanciare le politiche attive del lavoro del nostro Paese, anche allo scopo di scongiurare i rischi di immediate e gravi ripercussioni occupazionali derivanti dalla fine del blocco dei licenziamenti; quali iniziative voglia intraprendere per promuovere il reinserimento lavorativo e l'innalzamento dei livelli occupazionali, anche alla luce degli scarsi risultati ottenuti negli ultimi anni.

e il contestuale blocco dei licenziamenti e l'individuazione di ulteriori strumenti di sostegno al reddito per i soggetti che non si era riusciti a raggiungere con gli interventi precedenti, il Governo ha inteso garantire una rete di protezione il più possibile inclusiva ed equa, che facesse da argine all'impatto devastante della pandemia, in continuità - io credo - con alcune scelte precedentemente assunte. Fin dal mio insediamento, ho cercato di coniugare le misure straordinarie di protezione dei lavoratori, con l'avvio di due riforme strutturali che ritengo prioritarie: quella degli ammortizzatori sociali e quella delle politiche attive. Dobbiamo dare ammortizzatori a milioni di lavoratori che oggi non li hanno. E dobbiamo agire sulle competenze di base dei lavoratori più lontani dal mondo del lavoro e fornire una formazione più avanzata anche per quei lavoratori più qualificati che comunque potrebbero trovarsi in una situazione di transizione nei prossimi mesi e avranno bisogno di un accompagnamento della ricollocazione; ciò anche perché molti indicatori ci dicono che non è detto che la ripresa riprodurrà i posti di lavoro che si sono determinati negli stessi ambiti in cui sono venuti meno. Ritengo fondamentale adottare una visione organica, che racchiuda in un solo intervento l'insieme di queste iniziative, accompagnando così la trasformazione del mercato del lavoro e facilitando le transizioni occupazionali; migliorando l'occupabilità dei lavoratori e innalzando il livello delle tutele attraverso la formazione. Puntiamo quindi ad un pacchetto di misure adeguate per contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile, agendo sull'intero percorso che dalle misure di *welfare* che dalle misure di *welfare* può condurre al lavoro, e cioè fino al vero e proprio sbocco occupazionale. Per questo stiamo valutando misure specifiche da inserire anche nei prossimi provvedimenti d'urgenza che istituiscono luoghi di formazione all'interno dei contesti produttivi. Introduciamo così un intervento innovativo di politica attiva basato sul partenariato pubblico-privato per mettere in connessione con continuità ed efficacia il sistema produttivo e la forza lavoro disponibile, attraverso lo sviluppo di servizi dedicati alla creazione di nuove opportunità. Anche sull'occupazione femminile stiamo già studiando specifiche proposte che agiscano innanzitutto sulle pari opportunità di lavoro per le donne, a partire dall'anticipazione della valutazione sull'impatto di genere, che già è contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il *gender procurement*, che stiamo cercando di inserire il prima possibile. Per scongiurare i rischi dei prossimi mesi, quando lo sblocco dei licenziamenti sarà suscettibile di determinare gravi ripercussioni occupazionali, stiamo valutando alcune misure volte ad incentivare il reinserimento lavorativo e l'innalzamento dei livelli occupazionali. Si tratta dell'introduzione di nuovi strumenti che garantiscono alle imprese la necessaria flessibilità nella delicata fase della ripartenza e ai lavoratori un percorso contestuale di formazione, di adeguamento mirato delle competenze e di inserimento lavorativo, in grado di accompagnarli nelle transizioni occupazionali verso un impiego stabile. Credo poi che sia urgente, urgentissimo, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, iniziare a fare una mappatura dell'andamento dei diversi settori, perché la ripresa non è uguale, non sarà uguale da tutte le parti e dentro gli stessi settori ci sarà un'articolazione diversa e un rimbalzo diverso. Il monitoraggio è quindi molto importante anche perché continuare a utilizzare strumenti uguali per situazioni diverse non sempre è il meglio che si possa fare in questa fase storica.

situazione della Whirpool in tale città. Lei sa che la Whirpool nonostante abbia presentato i risultati del primo trimestre in Europa, riferendo una crescita doppia nei ricavi, ha comunque deciso di chiudere i battenti a Napoli, lasciando così a piedi, a casa, 330 lavoratori. Signor Ministro, lei sa che la situazione della Whirpool, tra l'altro, è simile a quelle di altre aziende e di altri grossi gruppi del Sud, che tra poco chiuderanno, lasciando a casa migliaia di operai. Mi rendo conto che, dati i tempi contingentati previsti dal Regolamento, non posso pretendere da lei una risposta, ma almeno vorrei da lei un impegno, che non sia formale, ma sostanziale, affinché finalmente queste importanti questioni siano affrontate dal suo Ministero e all'interno del Governo, alla luce anche dei notevoli finanziamenti all'interno del PNRR per il Sud. Lo dico da napoletano, da campano, da uomo del Sud, ma soprattutto - mi permetta, Ministro, da italiano: se non riparte il Mezzogiorno, non riparte l'Italia.

signor Ministro, la tutela e la promozione del lavoro sono per noi di Fratelli d'Italia un impegno politico quasi esistenziale e rappresentano, almeno per un Ministro della Repubblica e soprattutto per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un dovere. Vogliamo interrogarla sul tema del reddito di cittadinanza. Difendere il lavoro, per chi ha una cultura liberale come me, vuol dire innanzitutto investire nel lavoro, promuovere le le imprese che assumono e difendere quelle imprese - penso alla Silvelox del Trentino-Alto Adige o all'ex Embraco del Piemonte che invece vedono i propri lavoratori a rischio di perdere il posto per delle complicazioni giuridiche inutili, che esistono purtroppo nel nostro ordinamento e anche per posizioni non accettabili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ecco questo significa difendere il lavoro ed i lavoratori. Posso comprendere - so che lei non si offenderà, signor Ministro - che la sua cultura sia diversa dalla mia; la sua matrice marxista certamente ha una visione differente dalla mia visione liberale. Credo però che dovremmo e potremmo convenire, signor Ministro, che il reddito di cittadinanza si è dimostrato una mera misura assistenziale. Non lo dice Fratelli d'Italia, lo dicono i dati dell'Agenzia nazionale 1.650.000 percettori del reddito di cittadinanza, 423 assegni di ricollocazione attiva, zero posti di lavoro creati. Questi sono numeri che testimoniano il fallimento del reddito di cittadinanza come promozione del lavoro, come creazione di posti di lavoro;

Prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, la proroga degli scandalosi incarichi ANPAL e quindi - ecco il per i *navigator* nei concorsi pubblici: su 11.000 posti pubblici che andranno a concorso, ne avremo di fatto più della metà già assegnati o quasi. Signor Ministro, è su questo che la voglio interrogare interrogare e chiedere un riscontro preciso: non ritiene che la meritocrazia sia sacrificata ai privilegi degli amici e ai privilegi di qualcuno, e quindi che sia veramente una perdita grave per le potenzialità del nostro sistema Paese? Non è accettabile che il decreto-legge sostegni, il provvedimento che dovrebbe aiutare le nostre imprese e quindi i nostri lavoratori,

Bertoldi, la ringrazio della domanda. Non sono assolutamente offeso se sottolinea che la sua cultura politica è diversa dalla mia e non posso che compiacermi che la cultura liberale si sia così ampiamente diffusa. *(Applausi)*. Quello che ritengo invece giusto sottolineare è che il rispetto della verità ci dice che, nell'ambito del decreto-legge sostegni, non c'è nessuna proroga degli incarichi dell'ANPAL, che non sono soggetti a *spoil system*,

Questa vicenda ci consiglierebbe di non utilizzare più termini inglesi per definire delle funzioni che si esercitano in questo Paese perché, più che una definizione, rischiano di diventare uno stigma. Non c'è nessun privilegio né lede le pari opportunità di accesso alle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, atteso che gli stessi devono sostenere e superare le prove degli eventuali concorsi a cui volessero partecipare, come peraltro è già avvenuto in alcune Regioni in cui hanno partecipato. La valutazione favorevole delle pregresse esperienze - quando ci sono state - nella selezione sostenuta corrisponde a un principio già ampiamente utilizzato nella pubblica amministrazione e peraltro confermato dalla recente normativa introdotta dal collega Brunetta. Ritengo quindi che l'attività dei *navigator* vada considerata come una delle facoltà e delle conoscenze acquisite di chi parteciperà al concorso, in un'ottica che può concorrere al rafforzamento dei centri dell'impiego. Mi auguro che la stessa attenzione dedicata a questo tema sia rivolta anche ai gravi ritardi che ancora purtroppo caratterizzano il processo di assunzione degli 11.000 posti previsti all'interno dei centri per l'impiego, con risorse già stanziate, e che passano attraverso una serie di piani e bandi realizzati dalle Regioni che considero assolutamente essenziali per realizzare nel nostro Paese un sistema politiche attive del lavoro che non può che vedere protagonisti i soggetti privati, ma anche una rete pubblica che deve essere messa nelle condizioni di sostenere adeguatamente questa sfida. Il completamento in tempi rapidi di questo processo credo sia fondamentale perché le strutture territoriali siano in grado di

che valutare la capacità di realizzare politiche attive del lavoro nell'ambito di una pandemia sia abbastanza complicato. Credo che oggettivamente il reddito di cittadinanza sia servito a far fronte a a quella che rischiava di essere un'esplosione della povertà assoluta all'interno del nostro Paese. Valutiamolo per questo, e quando avremo un sistema delle politiche attive valuteremo anche cosa funziona e cosa non funziona. Credo che le due sfere vadano maggiormente distinte, però penso che sia giusto testarlo anche alla luce di un quadro

signor Ministro, non sono particolarmente soddisfatto - lo potrà capire - anche se ho considerato una certa difficoltà da parte sua, quale rappresentante del Governo, nel giustificare questo titolo di preferenza verso i *navigator* nei concorsi pubblici che, come recita l'articolo 18 del decreto-legge sostegni, esiste. Noi non lo condividiamo, perché - ribadisco - la meritocrazia deve prevalere su tutto; non vogliamo privilegi

molto importante, ossia l'ipotesi di introdurre un salario minimo legale. Siamo partiti da alcuni disegni di legge depositati da molto tempo in Senato e anche grazie all'impulso di chi l'ha preceduta al Ministero. Poi, naturalmente, la pandemia ha mandato a gambe all'aria l'agenda politica. Tuttavia, signor Ministro, ritengo non vi sia un solo motivo

perché si sta occupando di capire che cosa accadrà il minuto dopo la rimozione del blocco dei licenziamenti, in relazione soprattutto alla riforma degli ammortizzatori sociali cui ha fatto riferimento. Tuttavia, non è meno mortificante

che riguarda le iniziative che si intendono adottare per migliorare l'adeguatezza dei salari e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. È di qualche giorno fa la notizia che il nostro Paese ha avuto tra le più forti perdite del potere d'acquisto dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. Il tema è di primaria importanza, in particolar modo nel momento attuale, perché la pandemia ha duramente colpito l'economia europea e risulta essenziale assicurare salari che siano adeguati, sufficienti a garantire ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della nostra Costituzione. La determinazione di una soglia di salario minimo favorirebbe la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le diseguaglianze anche in termini di *gender pay gap*. Su questo tema ritengo sia opportuno stare dentro al quadro che si sta definendo a livello europeo. La proposta di direttiva della Commissione contiene regole volte a rendere più efficaci e uniformi i sistemi adottati dai Paesi dell'Unione europea, perseguendo l'obiettivo comune di rendere accessibile a tutti i lavoratori la tutela di un trattamento salariale minimo e rafforzando ed estendendo la copertura della contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Questo quadro di riferimento definirà alcuni principi e criteri ordinatori ai quali attenersi, che ci consentiranno di giungere a un'eventuale individuazione normativa del salario minimo e soprattutto di chiarire e risolvere la questione del rapporto tra rappresentanza sindacale e salario minimo, che nel nostro Paese costituisce una difficoltà storica. Occorre infatti potenziare la contrattazione collettiva attraverso un intervento legislativo in materia di rappresentatività sindacale, che credo sia necessario a salvaguardare il salario minimo da fenomeni distorsivi e a tutelare il più possibile i lavoratori. La direttiva ci darà un riferimento su come agire e come intervenire in questa direzione. Sarà quindi un necessario punto di riferimento che può implementare e rafforzare un principio di democrazia economico, che considero non solo auspicabile, ma anche necessario. Signor Ministro, le sue parole dicono evidentemente non solo della sua sensibilità, ma anche della volontà di procedere proprio sulla strada dell'introduzione di una soglia minima salariale. Penso che abbiamo bisogno di farlo per lasciarci alle spalle almeno due dibattiti, o comunque il modo con cui li abbiamo affrontati in passato. Mi riferisco anzitutto a quello sulle politiche industriali, tanto più alla luce di quanto accaduto in questi mesi. Non si può immaginare di entrare nel mondo nuovo pensando che si possono aiutare le imprese non stando sul terreno della qualità e dell'innovazione, ma immaginando una pressione verso il basso dei salari. Ecco, questa è una discussione vecchia, superata, che dobbiamo lasciare alle nostre spalle. Ce n'è un'altra, che è echeggiata persino in quest'Aula quando l'abbiamo affrontata, e cioè quella che mette in contrapposizione gli strumenti a cui lei ha fatto riferimento (sostegno al reddito, reddito di cittadinanza, forme universalistiche di sostegno al reddito) alla questione

perché queste spingono soprattutto i giovani a poltrire sui loro divani e li disincentivano alla ricerca di un lavoro. Infatti, quando i giovani confrontano il lavoro che hanno fuori e il reddito che ricevono, preferiscono il secondo. Ecco, semmai fosse vera questa tesi, allora vuol dire che bisogna alzare i salari e che quindi il problema è quello salariale che questo Paese deve affrontare anche introducendo una soglia minima legale. La ringrazio per la risposta e soprattutto per quello che potrà fare.

l'emergenza epidemiologica, infatti, sta compromettendo importanti settori economici del nostro Paese che, prima della pandemia, erano in forte crescita (ad esempio il settore del turismo) e sta determinando gravissime conseguenze occupazionali con rapporti a termine in forte riduzione, senza un'adeguata crescita dei contratti a tempo indeterminato; secondo i più recenti dati, a dicembre 2020 risultavano quasi 393.000 contratti a tempo determinato in meno rispetto a un anno prima, considerando gli occupati, mentre per quanto concerne quelli di nuova attivazione nel corso del 2020 si sono registrati 1,4 milioni di contratti in meno rispetto al 2019; il decreto-legge n. 87, noto come decreto "dignità" ed improntato al ragionevole obiettivo di favorire la costituzione di rapporti di lavoro sempre più stabili, era però pensato per un assetto socio-economico del tutto differente da quello a pandemia in corso. Nel decreto n. 34 del maggio 2020, in ragione dell'emergenza pandemica, avevamo previsto la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti a tempo determinato, in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19. A sua volta, l'articolo 17 del decreto-legge n. 41 del marzo di quest'anno, prevede che fino al 31 dicembre 2021 i contratti a tempo determinato possano essere rinnovati o prorogati per massimo dodici e per una sola volta, anche in assenza della condizionalità presente a normativa vigente, ferma restando la durata complessiva massima di Le misure sinora adottate non sono però sufficienti, in quanto l'emergenza in corso impone una riflessione più ampia sull'attuale assetto normativo dei rapporti di lavoro. In un momento di grave crisi economica, è indispensabile consentire la prosecuzione dei contratti a termine, *in primis* perché le imprese non riescono a stabilizzare, vista l'incertezza economica. Si rischia dunque di non offrire continuità occupazionale a questi lavoratori di disperdere delle professionalità eccellenti. La proroga consentirebbe dunque di mantenere un legame tra lavoratori e impresa. Alla luce di tutto questo, signor Ministro, le chiediamo quali iniziative intenda adottare da subito, in merito

sociali*. Signor Presidente, come è noto e come è stato ricordato, nel decreto-legge sostegni abbiamo prorogato la sospensione delle causali dei contratti a termine, in coerenza con la proroga delle altre misure emergenziali che sono state adottate a protezione dell'occupazione, a fronte del protrarsi del quadro emergenziale e della sospensione delle attività produttive. Sono consapevole che le imprese chiedono la revisione del decreto-legge dignità per alleggerire i limiti posti dalla contrattazione a termine e garantire condizioni di maggiore flessibilità che possano essere di stimolo alla ripartenza. In un'ottica di medio e lungo periodo certamente occorre soffermarsi sulla disciplina concernente il mercato del lavoro e le relative tipologie contrattuali. Bisognerebbe però analizzare con attenzione i dati sul processo di stabilizzazione dei contratti a termine, tenendo anche conto dell'elemento distorsivo della pandemia. che bisogna respingere ogni tentazione di ritorno alla precarizzazione e per questo motivo non credo sia opportuno pensare - insisto molto su questo concetto - a strumenti che siano validi per tutti gli ambiti e che agiscano nello stesso modo. La crisi pandemica, rispetto alle crisi precedenti, ha una sostanziale differenza, perché ha avuto un impatto molto eterogeneo sui diversi settori produttivi. Se è giustificata l'impossibilità di stabilizzare in settori che sono fortemente colpiti dal virus, lo è meno in settori che, invece, nel corso di questi mesi hanno continuato a crescere e sono stati in una condizione

parti sociali - di come si differenzia, di come si creano dei tavoli di settore, di come si porta il dialogo sociale a livello territoriale, perché considero che questo sia l'unico modo di distinguere. oggi che ci inventiamo un nuovo contratto, che ha caratteristiche di maggiore flessibilità, valido in tutti i settori, significa in alcuni casi probabilmente fare troppo poco e in altri indurre un processo di precarizzazione, che in questo momento non è auspicabile. Quindi penso che dovremmo studiare, per l'auspicato rimbalzo, dei "vestiti" fatti in qualche modo su misura per i diversi comparti. Questo è lo sforzo che credo dovremmo fare nelle prossime settimane, sperando che il dialogo sociale vada anche un po' oltre il tema del blocco dei licenziamenti o della data relativa a tale blocco, che pure è sicuramente una questione importante, ma assuma anche il tema di come si costruiscono strumenti che tengano conto delle differenze territoriali e di settore. *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, prendiamo atto di questa sua risposta puntuale. Colgo l'occasione anche per segnalarle un altro aspetto importante, che alla Lega-Salvini Premier sta particolarmente a cuore. Quasi il 90 per cento dei lavoratori agricoli è impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, in cui il reddito dipende dal numero

impiegati nelle imprese agricole rischiano di rimanere senza giornate lavorative nel corso del 2021. Noi della Lega abbiamo due proposte: quella di estendere la cassa integrazione in deroga

nel caso in cui lo debba richiedere l'azienda rispetto al lavoratore non funziona. Noi le chiediamo, signor Ministro, di ascoltare il grido di dolore e di solidarietà verso questi lavoratori.

vorrei esprimere la solidarietà mia e dei miei colleghi al gioielliere Mario Roggero, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Grinzane Cavour per la tragica rapina accaduta ieri. *(Applausi)*. Tre rapinatori hanno fatto irruzione nel suo negozio, lui, che già sei anni fa aveva subito una rapina violenta ed era stato selvaggiamente pestato mentre si trovava in negozio con la moglie e la figlia,

Signor Presidente, onorevole Ministro, con la legge di bilancio 2020 sono state istituite la commissione tecnica di studio sulla previdenza e l'assistenza e la commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni. Entrambe sono state prorogate al 31 dicembre 2021.

abbassando limite di unità lavorative in organico per accedere al beneficio da 1.000 a 250 unità; è stata altresì prorogata per il 2021 anche opzione donna, una misura che offre la possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro. del lavoro. Riteniamo necessario per il bene del Paese, soprattutto in questo momento molto particolare di crisi economica, continuare a promuovere misure come opzione donna e Ape sociale, rendere strutturale il contratto di espansione ed inserire nel quadro normativo la staffetta generazionale e l'istituto dell'isopensione, oltre che la pensione di garanzia per i giovani. Tenuto conto che in data 28 gennaio 2020 è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il decreto istitutivo del tavolo tecnico di studio sulle tematiche previdenziali, al quale è stato affidato il compito di definire le linee di indirizzo e gli interventi di riforma del sistema pensionistico, le chiediamo, onorevole Ministro: se intende portare avanti ed ultimare i lavori delle due commissioni richiamate in premessa; se intende inserire nel quadro normativo misure quali la staffetta generazionale, la pensione di garanzia per i giovani e l'isopensione; se intende istituire il tavolo sulle tematiche previdenziali, al fine di intervenire sul sistema pensionistico, considerato che la sperimentazione di quota 100 terminerà a dicembre 2021, oltre a confermare Ape sociale, contratto di espansione e opzione donna a decorrere dal gennaio 2022.

le commissioni tecniche che sono state istituite dall'articolo 1, dai commi 474 e 475, della legge del 27 dicembre 2019, il cui funzionamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, sono certamente organismi che considero essenziali per l'acquisizione di elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. L'insediamento di entrambe le commissioni è avvenuto nel mese di gennaio 2021, ma la transizione dal Governo Conte 2 al Governo Draghi ha determinato la necessità di acquisire le nuove designazioni dei rappresentanti dei vari Ministeri. Questa fase di sostanziale reinsediamento della commissione si è appena conclusa: con il decreto ministeriale n. 94 del 20 aprile 2021 si è provveduto a modificare la composizione della commissione sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale; ministeriale n. 101 del 27 aprile 2021 è stata modificata la composizione della commissione sulla gravosità delle occupazioni. La commissione sulla classificazione della spesa si è riunito proprio nella giornata di ieri, 28 aprile. Ad essa è stato assegnato il compito complesso in quanto la classificazione della spesa presuppone anche un'individuazione degli obiettivi che si vogliono perseguire e dei bisogni che si vogliono soddisfare. Pertanto, la riflessione sulla riforma pensionistica è già stata sostanzialmente riattivata sul piano tecnico e all'esito di queste settimane di approfondimento avremo gli elementi per valutare correttamente il peso e la composizione della spesa pensionistica e assistenziale presente e futura e per supportare congruamente le politiche pubbliche di sicurezza sociale. Con i risultati del lavoro delle Commissioni, si aprirà quindi un confronto con le parti sociali, con gli altri Ministeri interessati e in sede collegiale di Governo, al fine di individuare i percorsi adeguati per intervenire sul sistema pensionistico, anche al fine, tra l'altro, di valutare la permanenza di istituti previdenziali che consentono condizioni di flessibilità per categorie di soggetti svantaggiati e di individuare nuovi istituti di garanzia per i giovani, come auspicato dagli onorevoli interroganti. In ogni caso le proposte di intervento che saranno prossimamente individuate e condivise dovranno necessariamente essere orientate a garantire che il sistema sia sempre più aderente alle direttrici di fondo dell'equità generazionale, della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni aggiungo, a costo di essere monotono - alla fase del ciclo economico che si va determinando. Penso, ad esempio, che andrà agganciato a questo ragionamento un più intenso utilizzo dei contratti di solidarietà e dei contratti di espansione, che sono uno strumento che ha anche una ricaduta sul fronte previdenziale. Questa è la discussione che va fatta. Confesso - lo voglio dire con molta franchezza e me ne assumo la responsabilità che nelle prime settimane la mia attenzione è stata prevalentemente dedicata a chi il lavoro rischia di perderlo, senza sottovalutare il fatto che comunque c'è una legittima aspettativa di lavoratori che a fine anno vogliono sapere qual è il loro destino. tuttavia necessario, prima di tutto, raccogliere il lavoro che era stato fatto su questi due fronti: politiche attive e ammortizzatori sociali. Oggi possiamo dire che questo lavoro è stato riavviato e credo che ci siano anche le condizioni per aprire un confronto sul tema della previdenza.

Prendo atto che il Ministero ha riconvocato le due commissioni di studio sulla previdenza e assistenza e sulla gravosità dell'occupazione, che a mio avviso dovrebbero ultimare i lavori entro settembre di quest'anno, in modo da poter individuare alcuni interventi utili entro fine anno. Ribadisco l'importanza di ripristinare, nel più breve tempo possibile, il tavolo tecnico di studio sulle tecniche previdenziali al fine di definire gli interventi di riforma del sistema pensionistico. che, oltre alla proroga di opzione donna e Ape sociale, a rendere strutturale il contratto di espansione e alla possibilità di ottenere strumenti, quali la staffetta generazionale, l'isopensione e la pensione di garanzia per i giovani, sia necessario intervenire sul sistema pensionistico a partire dal 2022, inserendo già nella prossima legge di bilancio, considerato tra l'altro che quota 100 finirà la sperimentazione prevista entro dicembre di quest'anno.

Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, il cui elenco dei componenti è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna,

Signora Presidente, quanto emerge dall'inchiesta della testata "Fanpage.it" sul sottosegretario della Lega Claudio Durigon è grave e non ammette nessun tentennamento. È grave ed è necessario che venga chiarito, perché, occupando una posizione così apicale in un Dicastero delicato come quello dell'economia, in un momento in cui stanno arrivando ingenti fondi europei, non possiamo permetterci nessuna ombra. Inquietano questi intricati rapporti con l'UGL, inquieta che il bilancio di un sindacato non sia pubblico, anche se gestisce soldi dei lavoratori, inquietano i legami con imprenditori indagati dalla DDA; ed è inquietante l'affermazione che coinvolge la Guardia di finanza, che ci auguriamo essere totalmente falsa. Ma, se così fosse, saremmo parimenti in presenza di un Sottosegretario che si ammanta di vanagloria, tratteggiandosi come colui che è capace di condizionare i sistemi dello Stato. Allora, Presidente, occorre chiarire se siamo dinanzi a un millantatore che offende l'immagine e l'onorabilità del Governo o se ci sono fatti ignoti dietro ciò che è emerso da questa inchiesta, che meritano il vaglio dell'autorità giudiziaria. In ogni caso, le gravissime parole espresse dal Sottosegretario indicano una concezione assolutamente non compatibile con le funzioni di un esponente di Governo. *(Applausi)*. Per questo motivo, invitiamo il sottosegretario Claudio Durigon a rassegnare le proprie dimissioni.

il 29 giugno 2009 è una data tristemente nota per la strage ferroviaria di Viareggio, un disastro che si poteva e si doveva evitare, se si fosse investito in sicurezza e se non si fosse seguita la perversa logica del profitto, anziché quella della tutela della persona. Quella notte il fuoco avvolse un intero quartiere, bruciando trentatré persone, di cui tre bambini, che si pensavano al sicuro nelle loro case. Ciò che è successo in questi dodici anni è espressione del peggio della cialtroneria del nostro Paese: i tentativi di scaricare le responsabilità, la latitanza dello Stato, il depistare la verità, il tutelare i poteri forti invece che le vittime, la codardia e la mancanza di dignità nell'assumersi la responsabilità e nel chiedere scusa dinanzi a tanta sofferenza. L'allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti è stato condannato in primo e in secondo grado per reati gravissimi quali disastro ferroviario e omicidio plurimo colposo. Il cavalier Moretti - eh sì, perché poi, subito dopo la strage, l'allora presidente della Repubblica Napolitano lo insignì di tale onorificenza - invece di chiedere perdono o almeno scusa liquidò il disastro come uno spiacevole episodio, licenziando Riccardo Antonini, un ferroviere colpevole, a suo avviso, di aver fatto gratuitamente da consulente ai familiari delle vittime. Presidente, colleghe e colleghi, io come cittadino e ancor di più come parlamentare mi vergogno che ancora oggi a Moretti sia riconosciuto questo titolo, che non gli è stato revocato, come da anni chiediamo io, i miei colleghi, la città di Viareggio e tutti gli italiani che credono nella giustizia. questo non bastasse, ora ci giunge la notizia della nomina di Moretti a consigliere della partecipata statale PSC, nomina che magari lo porterà a cariche ancora più importanti. Questo è un ulteriore sfregio alle famiglie delle vittime, che a dodici anni da quel doloroso disastro, vedono ancora l'ex numero uno di FS ricoprire ruoli in società di pregio dello Stato. Io mi domando e vi domando: perché perché proprio lui? Perché non si ha un minimo di rispetto verso chi dovrà trascorre la propria vita rimpiangendo un proprio familiare? *(Applausi)*. Concludo dicendo che il cavalier Moretti non ha chiesto ancora scusa ai familiari delle vittime. Forse, stordito dalla sua tracotanza, non lo farà mai. signor Presidente, lo faccio io, con il cuore colmo di vergogna per rappresentare queste istituzioni che premiano i colpevoli e che, con questa nomina, uccidono ancora una volta quelle 33 persone innocenti per le quali, sia chiaro, non smetteremo mai e poi mai di chiedere giustizia.

per la questione appresa dagli organi di stampa in questi giorni relativa all'asserito ipotetico utilizzo dei voli di Stato da parte della presidente del Senato

per 124 volte, in undici mesi, dell'aereo di Stato: 97 volte nella tratta Venezia-Roma, cioè casa-ufficio della Presidente, e 6 ad agosto per la Sardegna. Esistono alcune norme al riguardo. Le ho studiate. Il decreto-legge n. 98 del 2011 dice che l'aereo in questione può essere usato certamente anche dalla Presidente del Senato, ma devono essere specificamente autorizzate le tratte e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Io chiedo allora come mai sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri non si trovi traccia di dette tratte. Quindi, o vengono smentite ma non mi risulta sia stata smentita la questione - oppure il sito è carente e, quindi, è stata violata la norma. C'è poi, ancora, la direttiva 23 settembre 2011, che stabilisce che l'utilizzo degli aerei di Stato può essere fatto soltanto per comprovate, imprevedibili e urgenti esigenze connesse alle funzioni e solo se c'è l'impossibilità di voli di linea e l'indisponibilità accertata di altre modalità di trasporto. Negli undici

che prevede la necessità di dettagliare le richieste, chiarendo esplicitamente i motivi e l'indisponibilità di altre tratte o altri voli. Allora, il punto è il seguente: qualora fosse confermata l'informazione e qualora le norme citate potrebbe essere prefigurabile il reato di peculato e comunque il danno erariale. Siccome la Presidenza del Senato rappresenta tutti noi, rappresenta quest'Assemblea, la questione deve essere chiarita, perché non è pensabile che i senatori della Repubblica siano rappresentati da una Presidenza che